Onorevoli colleghi, è con grande commozione che desidero ricordare, ad apertura della seduta odierna, Arrigo Boldrini, deceduto questa mattina, protagonista di straordinario valore politico e civile di alcune delle fasi drammatiche e cruciali della storia del nostro Paese, dalla Resistenza alla costruzione della Repubblica libera e democratica. A nome del Senato della Repubblica, e mio personale, voglio rinnovare pubblicamente ai suoi familiari il sincero e profondo cordoglio. Arrigo Boldrini, storico comandante partigiano, ha dato un contributo fondamentale alla lotta di liberazione contro il nazifascismo ed il suo coraggio, il suo altissimo entusiasmo per la giustizia e la libertà, le sue eccezionali capacità organizzative gli valsero la medaglia d'oro al valor militare. Per decenni alto dirigente del Partito comunista italiano e poi segretario dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, è stato uno dei nostri costituenti; anche grazie a lui, alla sua autentica passione politica, alla sua forte vocazione democratica, l'Italia ha potuto avere una Carta fondamentale, di cui domani celebreremo alla Camera il 60° anniversario, che rappresenta una delle pagine più alte del costituzionalismo europeo e pilastro vitale della nostra Repubblica. Deputato e senatore per molte legislature, Arrigo Boldrini ha sempre continuato le sue battaglie ideali per la promozione dei valori di libertà, di giustizia e di democrazia. La sua figura politica e il suo contributo rimangono per tutti noi un fondamento della Repubblica ed un esempio di amore civile per la nostra Patria, da riproporre costantemente alle giovani generazioni.

sulla figura di Arrigo Boldrini, del quale sono stato amico e compagno per oltre mezzo secolo. Della sua presenza nella Consulta, poi alla Camera e al Senato, ci ha parlato il Presidente. Al Parlamento Boldrini ha dedicato scrupolosamente il suo impegno politico e civile. All'italia ha donato il suo esempio. Arrigo Boldrini è stato un grande italiano, cresciuto nell'amore per la libertà, a cominciare dall'educazione ricevuta sin dall'infanzia dal padre, libertario romagnolo, ed alla causa della libertà ha dedicato la sua vita. Militare ed ufficiale nella Seconda guerra mondiale rientra, nell'agosto del 1943, nella città natale, in licenza di convalescenza dalla Jugoslavia (dove per un anno aveva comandato una compagnia di fanteria alle Bocche di Cattaro) e, alla folla riunita, alla notizia dell'armistizio, nella serata dell'8 settembre, Boldrini parla con grande passione e con forte determinazione, incitando all'unità nella lotta. La guarnigione dell'esercito, abbandonata dal comandante, si sfascia; comincia subito l'addestramento per il passaggio alla guerriglia. Nominato comandante - il comandante Bulow - della piazza di Ravenna, quando l'VIII Armata inglese si attesta attorno a Cervia, salpa dal litorale di Porto Corsini in barca a remi, attraccando a Milano Marittima il 18 novembre. Prende contatto con il comando del 1° Corpo d'armata canadese e concorda il piano per un'operazione congiunta tra partigiani e forze alleate per la liberazione della città. I partigiani cominciano a muoversi in diverse colonne, per dare inizio a quella che fu chiamata la «battaglia delle Valli» a nord di Ravenna. Al suo comando, una formazione di circa 700 uomini si appresta ad attaccare i capisaldi nemici disseminati fra gli acquitrini; riesce a superare le difese tedesche, nonostante lo sbarramento dei carri armati e dell'artiglieria pesante. Ferito, continua a combattere, lasciando stupiti anche gli alleati inglesi per il suo valore. La battaglia si conclude il 6 dicembre. Ravenna è libera. E da Ravenna Boldrini continua con i partigiani, a fianco degli alleati, la guerra di liberazione verso il Nord. Il 4 febbraio 1945, a guerra conclusa, a Ravenna, il generale Richard McCreery, comandante in capo dell'VIII Armata, decorerà di medaglia d'oro al valor militare Arrigo Boldrini in quella stessa Piazza Garibaldi dove, nella serata dell'8 settembre, egli aveva incitato la folla al combattimento contro nazisti e fascisti. Alla fine della guerra, Boldrini diverrà presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, animatore dell'intesa fra tutte le associazioni partigiane e combattentistiche e, più recentemente, anche presidente della Fondazione

grazie al quale si è riusciti allora a realizzare l'unità delle diverse formazioni militari, di tutte le brigate che facevano capo, distintamente, a comunisti, socialisti, cattolici, repubblicani, liberali, monarchici. Unico caso in Europa. Neppure in Jugoslavia, dove la Resistenza fu imponente, si era riusciti a realizzare l'unità di tutte le formazioni militari. I vincoli di solidarietà cementati nel corso della guerra fra quegli uomini (Ferruccio Parri, Luigi Longo, Enrico Mattei, Riccardo Lombardi, Sandro Pertini, Giorgio Amendola) rimarranno sempre vivi. Straordinari, persino emblematici, i rapporti di fraterna amicizia tra i due grandi ravennati: il comunista Boldrini e il democristiano Benigno Zaccagnini, il partigiano "Tommaso Moro". Una storia parallela cominciata nella canonica di Piangipane, paese ad una decina di chilometri da Ravenna. Amici sino alla fine. Avevano fatto un patto, dopo la guerra: chi fosse sopravvissuto avrebbe fatto all'altro il discorso al funerale. E così è stato. Fu Boldrini a tenere l'orazione funebre per l'indimenticabile segretario della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini nel novembre del 1989. Ricordare Boldrini, onorevoli colleghi, ricordare quegli uomini che ci hanno indicato l'esempio dell'unità e che l'hanno saputa costruire per la libertà, per il rinnovamento democratico dell'Italia, per il progresso sociale è oggi per tutti noi - credo - ammonimento severo. In questa nostra Italia, scossa in questi tempi da tante bufere politiche, sociali, civili, è questo l'impegno che mi sento qui di esprimere, io, partigiano come loro, oggi unico appartenente al Corpo volontari della libertà in quest'Aula, a voi tutti. Per la Repubblica, per l'Italia democratica.

Presidente, ero amico ed avversario di Arrigo Boldrini. L'ho conosciuto, ci siamo incontrati, abbiamo parlato tante volte e, nella differenza di valutazione, confrontato le nostre opinioni. Sarà consentito ad un vecchio liberale di parlar bene di un vecchio comunista che non c'è più. È stato detto che, nel nome della libertà, sono stati compiuti e si sono verificati grandi affratellamenti e, accanto ai partigiani poco fa ricordati, voglio anche ricordare il comandante Mauri che, nelle valli cuneesi, tenne alto il prestigio di quello che doveva essere un valore che una monarchia lontana non aveva saputo a suo tempo cogliere. I liberali hanno partecipato tanto al Comitato di liberazione nazionale per l'Alta Italia quanto alle responsabilità conseguenti, fino a quando sono state ritenute coerenti con una linea politica comune, in una valutazione di interessi e di valori. Vorrei unirmi a quanto detto poco fa dal senatore Cossutta perché capisco che, in certi momenti, i ricordi delle persone che hanno saputo affrontare i rischi, quando vi erano davvero, costituisce un esempio ed un valore che non può essere facilmente dimenticato. Sarebbe bene che, indipendentemente dal colore politico, si ricordassero coloro che per la libertà hanno fatto dei sacrifici, compreso quello di se stessi, affrontando il rischio che ciò comportava per la propria vita, per amore dell'Italia e della libertà. Presidente, colleghe e colleghi, lasciatemi aggiungere soltanto un piccolo ricordo personale, dal momento che ho fatto parte della Resistenza. Quando all'ANPI,

il Gruppo UDC non annovera Boldrini tra i personaggi di appartenenza di partito. Ritiene importante l'esperienza complessiva che Boldrini ha rappresentato nel nostro Paese, alla quale hanno partecipato tutti quelli di noi che hanno concorso a volere la libertà nel nostro Paese ed a garantirla dopo la fine della Seconda guerra mondiale. In questo senso è un ricordo molto positivo anche per noi.

figura di partigiano, protagonista della lotta di Liberazione, costituente, a lungo parlamentare della Repubblica che, con la sua azione nell'immediato dopoguerra e nelle fasi successive, ha sicuramente dato lustro ai valori fondanti della nostra Carta costituzionale che ella ha voluto prima ricordare.

della vita democratica e della Repubblica del nostro Paese. Mi fa piacere che esso sia stato caratterizzato da una convergente valutazione nell'Aula del Senato. Credo che il migliore omaggio che si possa rendere

Come ho già manifestato in quella sede, personalmente non concordo sulla sospensione dei lavori del Senato, in assenza di una richiesta formale, da parte del Governo, di fiducia in quest'Aula e soprattutto di una specifica votazione.

fiducia che sicuramente è illegale nel momento in cui è stata posta nell'Aula della Camera. Credo che, avendo il tempo per poterlo fare, tale verifica debba essere compiuta. Diversamente, se a partire dalle Aule parlamentari

vie antistanti lo stadio Olimpico di Roma. Alcuni tifosi della squadra di calcio del Catania - e non si parla di scontri, ma di aggressione - sono stati aggrediti da tifosi giallorossi

hanno parlato di scontri tra tifosi. Il Ministero dell'interno, ad oggi, non ha adottato alcuna misura. L'Osservatorio del Viminale non ha detto qual è il risultato delle indagini che si stanno conducendo;

autorità e cattiva informazione. Ripeto: alcune televisioni, in particolare quella in cui è intervenuto il giornalista Maurizio Mosca, hanno parlato dei soliti siciliani e degli scontri tra tifosi, quando invece i tifosi rosso-azzurri del Catania sono stati impropriamente aggrediti, alle ore 11,30, così come

nell'occasione più rilevante, cioè in sede di comunicazioni dinanzi una delle Aule del nostro Parlamento, il Presidente del Consiglio ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia alla Camera dei deputati

Colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha preso atto della richiesta avanzata alla Presidenza del Senato dal Presidente del Consiglio di riferire nella giornata di giovedì, nell'Aula di Palazzo Madama, sulla situazione politica, comunicando altresì di voler porre, in esito al relativo dibattito, la questione di fiducia. Tale dibattito avrà quindi luogo giovedì pomeriggio con inizio alle ore 15. Ho chiesto al Presidente del Consiglio

Per la discussione generale sono state ripartite tra i Gruppi due ore e mezzo. Alle ore 17,45 inizierà la ripresa diretta televisiva, relativa sia alla replica del Presidente del Consiglio che alle dichiarazioni di voto.

In relazione alla situazione politico-istituzionale creatasi con la richiesta di fiducia alle Camere da parte del Presidente del Consiglio, l'Assemblea non darà corso all'esame degli argomenti previsti dall'ordine del giorno di oggi e dal calendario di questa settimana. Analogamente, le sedute delle Commissioni non avranno luogo. Resta confermata per domani, alle ore 11, presso la Camera dei deputati, la cerimonia celebrativa del sessantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana. Onorevoli colleghi, il Ministro *ad interim* della giustizia ha trasmesso in data odierna, ai sensi dell'articolo 86 della legge sull'ordinamento giudiziario, la Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007, nel testo già comunicato il 16 gennaio scorso alla Camera dei deputati.

perché tutti siamo capaci di fare i conti. Pertanto, vi può essere il dubbio che il blocco dei lavori sia stabilito al fine di evitare la trappola della mozione di sfiducia individuale. Quindi, delle due l'una: o prima di domani pomeriggio arriva la richiesta formale del Presidente del Consiglio, suffragata dalla decisione del Consiglio dei ministri, così come vuole la legge,